Onorevoli colleghi, la Presidenza, alla luce dell'andamento dei lavori e nell'interesse della discussione sul disegno di legge sulla durata dei processi, preannunciato alla Conferenza dei Capigruppo la propria intenzione di procedere, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, all'accantonamento e al rinvio alla Commissione giustizia degli emendamenti presentati lunedì sera dal relatore e dei relativi articoli. Pertanto, la Commissione giustizia è immediatamente autorizzata a convocarsi. Alla luce di tale decisione, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha convenuto che l'Aula tornerà a riunirsi per il seguito della discussione del provvedimento questo pomeriggio alle ore 17, fino alle ore 21. L'esame proseguirà poi domani mattina, secondo gli orari già stabiliti, e la prossima settimana, martedì 19 gennaio, in un'ulteriore seduta da convocare alle ore 11, fino alle ore 13,30, nonché nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 16 alle ore 21, e mercoledì 20 dalle ore 9,30. Alle ore 12 di mercoledì inizieranno le dichiarazioni di voto finali con trasmissione diretta televisiva. Pertanto, il voto finale avrà luogo intorno alle ore 13 di mercoledì 20 gennaio. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre proceduto ad una nuova ripartizione dei tempi, assegnando - in aggiunta ai tempi residui - un'ora al Gruppo del Partito Democratico, 30 minuti al Gruppo dell'Italia dei Valori, 25 minuti al Gruppo UDC, SVP e Autonomie e 18 minuti al Gruppo Misto.